relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, essendo un mero succedaneo non posso che rimettermi alla perspicua relazione che il presidente Vizzini ha licenziato. Sento, però, il dovere di integrare la relazione con alcune brevi note di condotta parlamentare. Credo infatti che proprio il presidente Vizzini meriti apprezzamento da parte di noi tutti, componenti della minoranza e della maggioranza,

anche sia dovere di chi rappresenta la maggioranza esprimere il proprio più schietto ringraziamento nei confronti della minoranza, la quale ha portato un contributo nitido un contributo nitido e di scandita qualità al provvedimento. Un grazie speciale va al Ministro, Renato Brunetta, che ha saputo seguire l'andamento di questo fondamentale articolato con una capacità di ascolto

Non voglio dunque far perdere tempo all'Aula con considerazioni che nulla potrebbero portare in termini di arricchimento alla relazione del presidente Vizzini; sento tuttavia il bisogno di sottolineare come la grande crisi che sta facendo facendo alluvionale irruzione nel nostro sistema economico e produttivo renda ancora più cruciale e decisivo il compito che viene affidato a questa legge sulla riforma del lavoro pubblico, anzitutto dal punto di vista quantitativo. Basti pensare come ormai sia acquisito alla letteratura internazionale il fatto che per ogni dieci punti di recuperata efficienza del lavoro pubblico si generino virtuosamente due punti di prodotto interno lordo. Ma anche laddove non volessimo accogliere questa prospettazione quantitativa, basterebbe un calcolo elementare: credo che portare a regime questa legge di riforma possa consentire di recuperare, ed è una stima prudente, un 20 per cento di produttività del fattore lavoro nel settore pubblico, il che banalmente in termini di *full time* *equivalent* significa, a regime, un risparmio di 25 miliardi di euro all'anno. quindi di grandezze straordinariamente importanti, così come è straordinariamente importante eliminare alcune distorsioni. È una distorsione grave quando tutti i carotaggi statistico-organizzativi confermano che vi è ben il 50 per cento delle risorse utilizzate dagli enti pubblici destinato non già all'erogazione di beni e servizi ai cittadini, ma alla vera sopravvivenza dell'apparecchiatura burocratica, che è stata invece istituita per soddisfare i bisogni dei cittadini. Il miglior privato comparabile, cioè il privato delle grandi organizzazioni, ha 15 contro 50; quindi, c'è un margine di recupero di 35 punti. Non è tollerabile, ad esempio, che il delta tra la media delle prestazioni degli enti pubblici e i *top* *performer* segni una differenza di circa 55 punti. Non è tollerabile che la produttività degli uffici del Sud sia esattamente la metà di quella degli uffici del Nord. Ma anche dal punto di vista qualitativo, proprio per la mappatura e la configurazione del sistema produttivo italiano, intessuto di imprese piccole e medie, il ruolo di sostegno, di supporto, di promozione, di conferimento di slancio amministrazione nei confronti di questo sistema è decisivo. Non possiamo consentirci un fardello, non possiamo consentirci una zavorra che proprio in questa fase drammaticamente difficile costituisca un inibitore della dinamica competitiva positiva delle nostre imprese. Il disegno di legge, così come è uscito dalla discussione, in sede di Comitato ristretto della Commissione, colpisce con forza il degenerativo modello di consociazione che ha tristemente segnato le relazioni industriali nel settore pubblico negli ultimi decenni. valorizza intensamente e densamente il merito, valorizza intensamente e densamente quella trasparenza che diventa vettore di efficienza e di qualità. È un grande provvedimento di modernizzazione del nostro Paese ed è quindi un autentico *booster* di capacità competitiva. Credo davvero, onorevoli colleghi, che si possa immaginare che qui si realizzi quel *reinventing* *government* che fu lo slogan di Bill Clinton e Al Gore nel 1994. Qui davvero stiamo reinventando il modo di governare, con efficienza, con qualità e con capacità di appropriazione del destino più vero del nostro Paese, la nostra pubblica amministrazione. *(Applausi Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

Noi invece siamo molto interessati e da sempre - lo abbiamo manifestato anche con le nostre proposte di legge - ad un vero discorso di riforma della pubblica amministrazione.

evidente rispetto ad altre esperienze. Questo perché la politica continua ancora a considerare la pubblica amministrazione un affare di burocrati e non un fattore di sviluppo del Paese. Le maggiori diseconomie del nostro Paese, soprattutto in alcune aree

sempre maggiori competenze rispetto al territorio, alle imprese e ai cittadini. Ecco perché noi, pur avendo lavorato molto seriamente sulla proposta di legge in discussione, abbiamo ritenuto insufficiente dal punto di vista riformatore la proposta portata dal ministro Brunetta - e dirò perché - e in alcuni punti addirittura negativa. Penso alla ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, sulla quale abbiamo

è che una vera riforma della pubblica amministrazione si fa centrando l'attenzione sul rapporto di lavoro, sulla contrattazione, sulle norme, sul ruolo della dirigenza pubblica, ma anche investendo

non saremo mai all'altezza dei tempi e delle sfide. Alcuni punti qualificanti sono stati introdotti: penso al tema della trasparenza e al rapporto con l'utenza. Non c'è dubbio che, poiché la pubblica amministrazione opera non in regime di concorrenza, uno degli elementi forti è quello della pressione sugli utenti, dell'attenzione ai risultati, di una valutazione seria. Tuttavia, a tale riguardo non ci ha convinto l'atteggiamento un po' retrodatato

che deve essere invece ancor più valorizzata non solo in questa legge, ma spero anche con altri eventuali provvedimenti e, soprattutto, con un'azione di più lunga durata sulla pubblica amministrazione. Il vero nodo, infatti, è che il datore di lavoro pubblico può, tra la legge e il contratto, introdurre numerosissime azioni di riforma e di riorganizzazione della pubblica amministrazione. È per questo che non abbiamo avuto dubbi ad affrontare il terreno dell'innovazione, perché sappiamo tutti che, nonostante vi siano state numerose riforme, da quella del decreto legislativo n. 29 del 1993 a le stesse norme, ma anche la stessa contrattazione hanno dato dal punto di vista dei risultati sicuramente molte ombre oltre che luci. Dunque, signor Ministro, su questo provvedimento faremo sentire ancora in quest'Aula la nostra proposta emendativa. Vogliamo continuare ad andare avanti sul terreno dell'innovazione, vogliamo sfidare questa maggioranza su una vera riforma della pubblica amministrazione e speriamo che si possa continuare davvero in questa direzione per l'interesse del Paese.

colleghi, nell'affrontare il problema dell'efficienza e della produttività delle nostre amministrazioni pubbliche, dobbiamo porci una domanda cruciale: che cosa è mancato nelle riforme Cassese e Bassanini degli anni privatizzato il rapporto di lavoro, omologando l'organizzazione e la struttura del rapporto di impiego pubblico a quelli delle aziende private,

l'impresa privata e la costringe all'efficienza: la "molla" del mercato. Quando la struttura produttiva opera nel mercato, la sua inefficienza è punita da un'opzione che è data ai suoi interlocutori, ai suoi clienti e agli utenti, quella che Albert Hirschman chiama l'opzione *exit*, la possibilità di andarsene con i propri piedi. Ma lo stesso Hirschman ci avverte che, laddove non è possibile dare all'utente e all'interlocutore della grande organizzazione l'opzione *exit*, è indispensabile che gli si dia almeno l'opzione *voice*, cioè la facoltà di protestare, interloquire e interferire con le decisioni dell'amministrazione, dell'organizzazione, dell'azienda in relazione ai suoi difetti. Nelle nostre amministrazioni pubbliche e nel loro rapporto con i cittadini fino ad oggi troppo sovente è mancata non solo, com'è inevitabile, l'opzione *exit*, ma anche l'opzione *voice*. E dove mancano sia l'opzione *exit* che l'opzione *voice* il rischio grave è del collasso dell'organizzazione. La nostra iniziativa legislativa su questo terreno, avviata nella legislatura precedente con la presentazione del disegno di legge

alla cittadinanza e agli utenti vedere con precisione che cosa accade, interloquire, protestare, chiedere conto del raggiungimento di obiettivi precisi, misurabili, controllabili.

dalla metà degli anni Settanta è diventata principio generale dell'ordinamento svedese e che negli anni successivi è stata fatta propria da tanti ordinamenti del Nord Europa, e il principio di misurazione e valutazione di efficienza e produttività. È doveroso riconoscere alla maggioranza, in particolare al relatore relatore su questi disegni di legge, senatore Carlo Vizzini, e al senatore Maurizio Castro il merito di aver subito colto l'importanza decisiva di questi principi e aver consentito che la Commissione affari costituzionali in sede redigente li introducesse nel testo unificato che è ora al nostro esame. Ne è uscito un testo nuovo rispetto a quelli sui quali è iniziato questo *iter* parlamentare, un testo nel quale questi due principi fondamentali assumono un carattere portante di grande rilievo. Certo, il testo ha ancora molti difetti, ma mi sembra che i principi innovativi che in esso sono stati introdotti in Commissione possano segnare una svolta importante nel nostro ordinamento delle amministrazioni pubbliche, ma anche nel loro funzionamento concreto, a una condizione ovviamente: che essi vengano interpretati correttamente in sede di esercizio della delega da parte del Governo. Su questo non mancheremo di vigilare con grande attenzione.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame quest'oggi ha visto un importante contributo dell'opposizione nel tentativo di apportare correttivi utili allo scopo di attenuare l'intento qualche volta "persecutorio" del ministro Brunetta nei confronti dei pubblici dipendenti, in un *mix* di dichiarazioni estemporanee e di provvedimenti legislativi assolutamente inadeguati. Abbiamo proposto emendamenti tesi a mettere al centro del provvedimento i cittadini utenti, con l'introduzione di un organo di controllo capace di verificare l'efficienza e la trasparenza dell'amministrazione pubblica. Un organo che, se messo in condizione di lavorare fuori da condizionamenti politici, potrà contribuire a determinare un rapporto più trasparente tra l'amministrazione e i cittadini. Rapporto che ancora oggi, in alcune parti del Paese e in alcune strutture dello Stato, lamenta un deficit di certezze dei tempi, di trasparenza procedurale, di valutazione dei risultati conseguiti dai singoli comparti della pubblica amministrazione.

non entra nel merito. Nonostante l'introduzione di questo nuovo organismo e le altre modifiche intervenute durante la discussione in Commissione, il provvedimento prevede un impianto ancora da discutere e alcune parti migliorative difficilmente saranno applicate, perché la prassi attuale del Governo va in tutt'altra direzione.

la ricerca di introdurre normative volte al rilascio di acconti contrattuali al di fuori della contrattazione collettiva; l'assoluta inadeguatezza degli stanziamenti a favore del rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici; la campagna politica contro la legge n. 104 del 1992 per l'assistenza a favore dei familiari in grave difficoltà;

Questi sono gli atti politici che il Governo ha messo in campo in questi mesi. Per tornare al provvedimento, le mie perplessità si riferiscono al mantenimento di uno spettro troppo esteso a favore delle deleghe previste nel provvedimento, soprattutto in ordine alla rilegifìcazione del rapporto di lavoro. Nonostante luci ed ombre, a partire dagli anni Novanta, con l'equiparazione tra lavoro pubblico e privato, si lavorò per tenere fuori la politica e le maggioranze politiche dalla regolazione dei rapporti di lavoro nell'amministrazione pubblica.

l'articolo introdotto sulla Corte dei conti, che ne rivede poteri e compiti, intervenendo in un ambito estremamente delicato, che rischia di mettere in discussione la terzietà della Corte. Si mina pesantemente l'autonomia della magistratura contabile e credo sia chiaro cosa possa significare questo scenario in tema di spesa pubblica. esempio, più corretto l'emendamento presentato dai colleghi Mauro e Bodega - il ruolo del sistema delle autonomie locali e della Regione, che, così com'è nel testo, non è ancora definito e andrebbe maggiormente chiarito alla luce del Titolo V della Costituzione e del probabile, anzi del certo federalismo fiscale.

l'ampiezza delle deleghe, non ad eliminarli completamente. Credo che dovremo vigilare attentamente sulla concreta trasformazione in atti delle deleghe introdotte dal provvedimento. l'amministrazione pubblica non è un terreno da arare dalla maggioranza di turno, né da quella attuale, né da quella precedente o da quella futura, ma un bene indissolubile del Paese, sia per la sua efficienza e trasparenza, sia nel non essere assoggettato alle maggioranze del momento.

L'altra questione su cui bisogna intervenire più decisamente, dopo averne tanto parlato, è l'effettivo decentramento delle funzioni con risorse adeguate del decentramento-federalismo). In realtà, questa è una parte di riforma limitata anche perché interviene sulle amministrazioni centrali, lasciando completamente da parte

siamo ancora ad indicare la necessità di fare di più, per esempio, in queste due direzioni. Sottolineo tre punti critici, a

che fare con vari tentativi di rendere più fluido e più efficiente il contributo delle persone nella pubblica amministrazione. Il primo punto riguarda il rapporto tra le fonti, cioè tra legge e contratto, nella regolazione dei rapporti; il secondo riguarda la gestione effettiva delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro in rapporto alla stessa contrattazione collettiva, quindi i temi della valutazione

molto criticabili e, per certi versi, anche regressive. Il fatto, ad esempio, di tornare ad una regolamentazione legislativa dei rapporti

generato una serie di prassi frammentate, disperse ed ingiustizie di trattamento, per non parlare dei clientelismi sostenuti da leggi e leggine. Per questo motivo negli ultimi anni si è sviluppato il metodo contrattuale.

sulle macrostrutture organizzative - come recita anche la Costituzione - ma è il contratto che deve essere riportato alla sua capacità di regolazione nei rapporti che riguardano le persone, il lavoro, le condizioni di lavoro. Questo è un punto che è stato chiarito, anche se nel testo sono presenti ancora delle sbavature. Naturalmente - e qui vengo al secondo punto la contrattazione non è immune da vizi, da possibili ritardi o distorsioni. Per questo abbiamo fortemente sottolineato la necessità di responsabilizzare gli attori, quindi sindacati e pubblica amministrazione, la dirigenza di cui si parlava prima. Non è riportando sotto l'usbergo della legge che si migliora il risultato: questo sembrerebbe questo sembrerebbe infatti dire che non abbiamo fiducia nella capacità della dirigenza, che è l'interlocutore principale, di gestire bene il rapporto, per cui gli mettiamo sopra una cappa legislativa. Noi riteniamo piuttosto che la valorizzazione e l'autonomia della dirigenza siano il modo vero perché una contrattazione si svolga secondo obiettivi di efficienza e giustizia, com'è nella logica del rapporto contrattuale. Per sostenere questo abbiamo valorizzato molto la valutazione dei risultati, fatta come si è cominciato a fare - non bene - da organismi indipendenti, secondo criteri

si tramuti in effettiva verificabilità ed oggettività delle valutazioni. Noi crediamo che questi due punti, che tra l'altro sono stati sostenuti nel disegno di legge che la nostra parte aveva proposto in Commissione in dialettica

vediamo che si realizza questa prima attività non è favorevole. Abbiamo la sensazione

Se riuscissimo a realizzare anche solo la metà di quanto scritto in queste pagine non avremmo solo una amministrazione efficiente, ma potremmo anche immaginare un cittadino meno diffidente e meno sospettoso nei confronti del servizio pubblico. Trasparenza, valutazione del pubblico impiego, valorizzazione del merito: questi sono i principi guida del disegno di legge in discussione. Tradotto in termini più divulgativi, significa aumentare lo stipendio del dipendente professionale e volenteroso e mandare a casa chi consegna un falso certificato medico per godersi la busta paga senza muovere un dito. Gli obiettivi sono nobilissimi, difficilmente non condivisibili, ma visti in 15 anni di mezze riforme, tavoli tecnici e retromarce, non possiamo farci prendere dall'entusiasmo. Si è già tentato di abbandonare gli automatismi nelle progressioni di carriera: formalmente scomparso il criterio della anzianità, è rientrato dalla finestra sotto forma di promozioni generalizzate, decise in sede di contrattazione integrativa. Per questo ritengo fondamentale aver sancito nel testo il principio della valorizzazione del merito mediante la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera. Aspetto però di capire come verrà attuato nel concreto. Ad oggi, non solo gli stipendi nel pubblico impiego sono cresciuti più che nel settore privato, ma i *manager* pubblici hanno anche visto le proprie retribuzioni aumentare del 50 per cento in cinque anni ed il numero stesso dei dirigenti è sensibilmente cresciuto senza alcun evidente impatto positivo sui servizi forniti. Se le code all'INPS non diminuiscono, perché i dirigenti dovrebbero percepire un *bonus* sullo stipendio?

E, se le amministrazioni sono prive di un sistema di valutazione adeguato, non possono essere erogati *bonus*. Qui comincia un altro problema: chi valuta il merito di dipendenti e dirigenti? Come si può quantificare il lavoro del dipendente pubblico? Prerequisito per ogni tipo di valutazione è la diffusione di una corretta informazione, quindi un'informatizzazione della pubblica amministrazione. Tutti i dipartimenti devono avere un sito *on line* dove rendono pubblici i loro dati. Funzioni, servizi offerti, personale, costi, numero dei dirigenti e loro retribuzione: senza trasparenza e senza Internet non ci sarebbe nulla da valutare. Per questo il calo del 3,2 per cento degli investimenti dell'amministrazione in *Investment Technology* non è un bel segnale. La strada da seguire è quella tracciata dal ministro Brunetta, che ha costretto mezza Italia a mettere *on line* l'elenco dei consulenti. Complimenti, Ministro, non so se riceverà il Nobel, ma sicuramente merita la gratitudine dell'Italia. Ammesso, dunque, che si riescano a fornire tutti i dati sulla base dei quali valutare il servizio pubblico, resta sul tavolo il secondo problema: chi giudica dipendenti e dirigenti? Il disegno di legge parla della possibilità che siano gli utenti ad esprimere un parere sul servizio fornito - e mi sembra un'ottima cosa e di un organismo centrale, costituito in posizione autonoma e indipendente. Siccome non ricordo autorità indipendenti che abbiano brillato per terzietà negli ultimi dieci anni, non vorrei stessimo creando un altro ente non indispensabile. Non sarà facile rispondere, per l'ennesima volta, alla stessa domanda: chi controlla i controllori? Credo che chiunque faccia parte di questa agenzia dovrebbe percepire uno stipendio simbolico di un euro e il resto del compenso dovrebbe essere stabilito in base ai risparmi che l'agenzia stessa produrrà all'interno del settore pubblico. Non so quanto potremmo risparmiare con una misura simile, ma sicuramente sarebbe un bel segnale per il Paese. Concludo affermando che il merito deve continuare ad essere la stella polare dell'azione di questa maggioranza. Non è più il tempo di promozioni di massa e di aumenti generalizzati. Pochi ricordano che il 30 per cento dei risparmi della riforma Gelmini verrà reinvestito sui professori. Speriamo non tutti allo stesso modo. Lo stesso discorso vale anche per l'università: dobbiamo andare avanti contro baronie e sprechi per poter investire risorse solo dove ne vale davvero la pena. Questo sarebbe, signor Ministro, davvero rivoluzionario.

Signor Presidente, fra gli elementi di novità che hanno caratterizzato questo avvio di legislatura - visto che è qualche mese che stiamo parlando della proposta del ministro Brunetta in particolare, l'attività di Governo, non possiamo non sottolineare la coraggiosa azione dello stesso Ministro. Un'azione diretta a scardinare una delle piaghe più largamente riconosciute e condivise, ma,

procede ad una velocità a scartamento ridotto rispetto ai ritmi progressivamente accelerati ai quali è costretta, ad esempio, l'impresa privata per reggere la concorrenza e stare sul mercato sul mercato. Quindi, è costante la lagnanza dei cittadini verso quella che, in estrema sintesi, si può chiamare la burocrazia. Si tratta di una sorta di «mostro tartaruga» che rallenta, quando non ferma, l'*iter* delle procedure, anche di quelle

o chi non ha provato il senso di impotenza davanti a sportelli scanditi da un'impalpabile apatia, magari incolonnati in una lunga fila di questuanti! Va sottolineato che spesso, spesso, per ottenere quello che ci spetta di diritto, sembra si debba chiedere un'attenzione particolare. Insomma, è il terreno di coltura di quel sistema di raccomandazioni che rappresenta anche il modo,

e lo spirito del suo "*j'accuse*" non può non essere sposato su tutta la linea, anche perché animato, non dal carattere punitivo, ma dalla volontà di ammodernare il Paese attraverso un più efficace ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione. È necessario riprendere i concetti meritocratici e ad essi affidarsi per promuovere chi è più capace e più si sacrifica: questa è una delle chiavi fondamentali per scardinare un sistema che, invece, procede su un terreno puramente anagrafico ed elegge l'anzianità a leva per promozioni ed avanzamenti di carriera. di carriera. Chi ha vissuto in prima persona un'esperienza amministrativa di una città, di un paese o di una Provincia e, quindi, l'evoluzione del concetto di

eletto direttamente dal popolo per avere più potere (nel senso etimologico del "poter fare"), ma poi spesso si trova in condizioni di sudditanza davanti al dirigente che lastrica il cammino di una pratica di ostacoli e di troppi "se" e "ma". enti locali, fino ad infilarci nell'imbuto degli apparati dello Stato che, per tradizione oltre che per nomea, sono elefantiaci, pletorici e spesso capaci di trasformare ogni procedimento in una sorta di fabbrica del duomo.

Noi crediamo che occorra procedere in fretta e che la gradualità serva soltanto se sono chiari gli obiettivi e definiti gli strumenti. corrispondono azioni che trovano nel Parlamento la loro piena legittimazione e quella spinta operativa capace di trasformare in atti concreti le buone intenzioni. La Lega Nord Padania ha proposto alcuni emendamenti che vogliono mirare alla migliore efficienza valorizzando la territorialità. È in questo senso che deve essere interpretata l'indicazione di concorsi che privilegino l'azione e l'appartenenza regionale e, magari, evitino quella transumanza dal Sud al Nord di intere falangi di pubblici operatori, in particolare di insegnanti, che talvolta - e non suoni come un discrimine aggrappati al loro accento d'origine faticano a farsi capire in una scuola dove imparare bene la lingua italiana è ancora primario rispetto alla pur sacrosanta necessità di studiare anche le lingue straniere. Certo, occorre anche dire che le retribuzioni prese a sé sono spesso non congrue al costo della vita, ma dobbiamo capire innanzitutto che proprio il costo della vita presenta sostanziali variabili legate alla latitudine e per ciò non è peregrina l'idea di salari calibrati sulle singole realtà. Credo che la funzione pubblica, o meglio la disfunzione pubblica, sia uno dei mali secolari di questo Paese: è figlia di un'Italia fondata sul clientelismo, sulle assunzioni indiscriminate come moltiplicatori del consenso politico. Va da sé che una riforma su questo terreno debba essere accompagnata da una analoga azione che impegna la classe politica a ridurre i parlamentari, a dar corso ai senati regionali e ad abolire gli enti inutili. Se si procede con fermezza e con coraggio su questo doppio binario, non solo si eviteranno sprechi e si smaschereranno i fannulloni, ma si avvierà quel processo di ammodernamento dello Stato che è una delle premesse fondamentali per tornare ad essere competitivi e salvaguardare le qualità di intelligenza e di professionalità che i nostri cittadini hanno nel loro codice genetico.

Signor Presidente, fa un certo effetto mettere a confronto i due testi, quello licenziato originariamente dal ministro Brunetta e quello che è oggi al Quello originario era figlio di una politica assolutamente aggressiva nei confronti dei dipendenti pubblici, protesa ad una pubblicità a poco prezzo nei confronti di una opinione pubblica che certamente in molti casi non ha di che rallegrarsi per il funzionamento della macchina pubblica nelle sue varie articolazioni, specie quando essa non gestisce servizi alla persona, non si occupa di sicurezza, quando non svolge funzioni essenziali per la tutela dell'incolumità e della salute delle persone, quando non si fa carico dei bisogni (penso al vastissimo e complesso mondo delle politiche sociali) sempre più complessi e crescenti nelle persone stesse, quando non prova a misurarsi, come fanno faticosamente e spesso in perfetta solitudine molte strutture pubbliche giorno per giorno, con la costruzione di un nuovo *welfare* in questo Paese, che è la vera, primaria esigenza economica e sociale del nostro Paese stesso. Un *welfare* post-fordista, un *welfare* che assume e fa propria la centralità della persona, cosa questa che produce profondi mutamenti nell'organizzazione dei servizi e del lavoro. Basti pensare a cosa significa declinare oggi la qualità delle prestazioni passando dai processi di integrazione dei servizi stessi, cosa significa assumere la centralità del territorio: vuol dire mettere in discussione organizzazione del lavoro, capacità, professionalità, strutture. Quello che voglio dire è che quella politica così punitiva nei confronti del lavoro pubblico assume la pubblica amministrazione come un tutt'uno, un indistinto, ma la realtà non è questa. La realtà è che quella che comunemente va sotto la definizione di pubblica amministrazione è una somma di cose assai diverse per origine, funzionamento e finalità concrete, per capacità effettiva di misurarsi con la complessità della nostra società e una politica che non sa discernere, che fa di tutta l'erba un fascio, non solo commette un errore di ingenerosità, ma fa del danno vero, allontana la parte più disponibile, le forze più impegnate in uno sforzo quotidiano e spesso solitario per il miglioramento della qualità del lavoro e delle prestazioni. E forse - e questa è una grande ed amara verità - una politica che si comporta così maschera la sua incapacità progettuale, gestionale e riformatrice delle pubbliche amministrazioni. È così che si spiega l'agitare populisticamente il tema dei fannulloni. Nessuno può difendere chi non lavora: chi non lavora va licenziato. Questo mi insegna la la storia del movimento sindacale, questo mi insegna la storia della Sinistra e del centrosinistra. Nessun cedimento su questo; ma questo è un problema, non è il problema. Forse diversa era, ed è tuttora, la storia di quella parte della politica, spesso trasversale negli schieramenti, che ha basato e basa il suo successo anche su uno scambio nefasto fra consenso e scarsa produttività della pubblica amministrazione e su quell'idea invasiva della politica che, anziché limitarsi al ruolo di indirizzo e di controllo che gli è proprio, pensa di gestire direttamente la macchina pubblica, mettendo così anche oggettivamente in crisi il ruolo e la funzione della dirigenza pubblica.

per qualsiasi ragionamento serio e davvero efficace di riforma della pubblica amministrazione. Si agita quindi il tema dei fannulloni per mascherare un'incapacità ed una non volontà vera di cambiamento ed innovazione. Non sarà stato certo un caso, infatti, che nel testo originario risulta non pervenuta la forza, la capacità, l'idea stessa del cambiamento e dell'innovazione, ma è esattamente di questo che ha bisogno il Paese e la funzione pubblica: è di questo che ha bisogno la pubblica amministrazione. invece ci siamo trovati in presenza di un testo il cui tasso d'innovazione consisteva nel voltare la testa all'indietro, guardando ad un tempo non proprio paradisiaco, i cui effetti pesano ancora addosso come dei macigni, riportando totalmente, e anche formalmente, sotto il cappello della politica, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro che con fatica dopo un lungo dibattito, nonché uno scontro culturale e politico in questo Paese, aveva trovato nella riforma D'Antona un punto avanzato di equilibrio e di unità con il mondo del lavoro privato. Per noi innovazione e cambiamento di riforma sono termini essenziali e vitali per ridisegnare le nuove pubbliche amministrazioni e questo ancor più oggi, in presenza di questa drammatica crisi, nella quale assai probabilmente si ridisegneranno parecchi profili del nostro sistema economico e sociale - e non solo del nostro, ma anche nel mondo - e che non può vedere assenti, o in una remissiva attesa della sua conclusione, le strutture della pubblica amministrazione. Per noi innovazione, cambiamento e riforma sono termini che hanno bisogno di uno sguardo proiettato in avanti e, soprattutto, di un grande protagonismo dei soggetti destinatari*in primis* di questi processi e quindi, innanzitutto, il mondo del lavoro pubblico,

lo dico a lei, signor Ministro, e a qualche suo collega di Governo che, invece, per una furia ideologica verso una parte del movimento sindacale, la CGIL in particolare, sta creando seri problemi all'interno del Paese.

nella gestione delle deleghe, di rispettare il dettato del Parlamento. Sappia, signor Ministro, che il nostro Gruppo parlamentare vigilerà dentro e fuori quest'Aula

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Italia dei Valori ha partecipato con forte intenzione e impegno alla discussione del provvedimento in esame ed ha tentato di dare contributi utili a smorzare quelli che considerava aspetti critici, che continuano a permanere e possono essere motivo interessante di discussione anche nel futuro. Ne considererò alcuni. L'impianto del provvedimento poggia sostanzialmente sull'idea di una prevalenza dei meriti del privato rispetto al pubblico; se ne sente un'eco diffusa: la prevalenza del mercato, la bontà del mercato. In realtà, sappiamo tutti che nella situazione italiana il mercato è tutt'altro che sciolto e libero dai condizionamenti della stessa politica e della rete di rapporti che si stendono tra l'economia e la politica. Basterebbe pensare a quanto la concorrenza in realtà manchi dall'economia italiana, a quanti settori di mercato protetto esistono. Basterebbe pensare al caso clamoroso dell'Alitalia, la Repubblica italiana si impegna ad aprire una voragine di debiti spaventosa per garantire ad alcuni privati l'esercizio

dunque in un contesto tutt'altro che sgombro di dubbi. In tale contesto, il provvedimento insiste più volte sul tentativo di determinare nuovi rapporti tra legislazione e contrattazione.

più volte il provvedimento insiste a suggerire che la legislazione possa e debba fissare limiti, addirittura anche quantitativi ed economici, allo spazio in cui si muove la contrattazione. terzo punto di criticità, che abbiamo più volte rilevato in tutti i nodi del testo, è una certa tendenza, che naturalmente non stupisce data la maggioranza che che ha elaborato il disegno di legge, ad attribuire potestà sempre crescenti ai vertici apicali. Insomma, un punto di vista politico, che poggia sostanzialmente sull'ideologia del presidenzialismo,

Su questo restano molti dubbi, perché i meccanismi di giudizio sulla validità del lavoro svolto, di critica della fannullonaggine e premio a chi lavora restano attribuiti, per adesso e fino a che non vi sarà l'agenzia,

colto dalla scuola media: il preside è stato identificato come un *manager* della scuola, ma i meccanismi di attribuzione di incremento dello stipendio si poggiano su fattori che poco hanno a che vedere con il merito dell'insegnamento. Nella scuola media superiore prendono stipendi più alti i docenti che dedicano un monte ore maggiore a quello dei colleghi in attività di tutoraggio, accompagnamento, presenza in biblioteca e così quando invece ciò che dovrebbe essere premiato è il merito della qualità dell'insegnamento. Qui c'è qualcosa che non torna, perché allora, senza volere, un provvedimento che dovrebbe incrementare i meriti sostanziali, in realtà ritorna su una dimensione quasi bassamente sindacale, se posso usare questo termine improprio, perché, alla fine, si calcolano unicamente le ore di lavoro senza guardare a cosa siano servite. Il problema della valutazione

ma - per entrare ancora una volta nel merito del valore del lavoro svolto - proprio in questi giorni abbiamo ricevuto moltissime lettere di dipendenti che aspiravano alla vicedirigenza e che si trovano conculcati nei loro diritti proprio perché la vicedirigenza verrebbe abolita. Infine, una osservazione di passaggio sulla logica materiale con cui i provvedimenti camminano in Parlamento e nella società: vi è una certa prevalenza -non stupisce dato lo strapotere mediatico della maggioranza - ad ad esercitare un ruolo promotore attraverso la linea degli annunci, a detrimento della specificità del lavoro delle Assemblee elettive. Questo provvedimento è partito

Questo significa adottare una logica che una volta, al tempo dell'assolutismo, si chiamava la regola del *motu proprio*. Il promotore dell'azione politica ad un certo punto esprime di getto delle intenzioni, le comunica alla platea alla platea della società e si suppone che questo debba significare l'apertura di una nuova fase di iniziativa politica. È qualcosa di intimamente contrastante con la logica, invece, del lavoro democratico delle Assemblee parlamentari.

fino forse alla estinzione il concetto serio e classico, che non dovrebbe mai essere messo in discussione, della tutela e delle garanzie per il lavoro. Oggi, parlare di tutela e garanzia per il lavoro è fuori moda. Sembra di non essere

È un inganno. delle garanzie e dei diritti dei lavoratori è un colpo inferto ad una tradizione nobile che anche la società più progressiva in senso dinamico non dovrebbe mai dimenticare. Se qualcuno si approfitta delle tutele e delle garanzie, non è questa una buona ragione per togliere le tutele e le garanzie. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, se potessi modificare la rubrica di questo provvedimento potremmo scrivere che la pubblica amministrazione è ad una svolta, naturalmente positiva.

per riavviare e corroborare i processi economici del nostro Paese. Una pubblica amministrazione, quindi, non più fattore di redistribuzione del reddito nazionale con il fine di dare un posto a qualcuno, ma fattore di erogazione dei servizi e per dare cittadinanza a a quei diritti sociali che fanno sì che i cittadini siano più uguali nel momento in cui sono più elevate le differenze economiche e finanziarie: omogeneità di funzioni ed omogeneità di trattamento nella pubblica amministrazione. Soprattutto, si supera il percorso di una pubblica amministrazione che trae origine sin dalle prime leggi dell'Unità d'Italia. Vittorio Emanuele Orlando, nel suo primo trattato sulla pubblica amministrazione, aveva definito l'impiego alle dipendenze dello Stato come il potere dell'uomo sull'uomo. con questa legge noi prevediamo un criterio direttivo preciso, per cui coloro i quali sono alle dipendenze della pubblica amministrazione realizzano il bene pubblico

onore e che servire il Paese costituisce un privilegio per coloro i quali sono alle dipendenze della pubblica amministrazione e non soltanto un fattore di impiego e di occupazione. Trent'anni fa, in questa Aula del Parlamento, giunse il rapporto della commissione Coppi, che aveva indagato a lungo sulla cosiddetta giungla delle retribuzioni: 4,5 milioni di di pubblici dipendenti governati da logiche ordinamentali diametralmente opposte, ma soprattutto con trattamenti differenziati, non in relazione alle prestazioni, alle qualità ed alle responsabilità responsabilità ma per l'effetto e l'incidenza di una molteplicità di strumenti normativi, che naturalmente determinavano conflitti e soprattutto sproporzione e lesione di un precetto fondamentale, l'articolo 36 della Costituzione. questo è uno dei criteri direttivi di questa legge delega: proporzione delle retribuzioni dei trattamenti e delle funzioni alla qualità e quantità del lavoro prestato. Credo, signor Ministro, che da questa legge piuttosto importante il legislatore delegato non possa allontanarsi molto, perché tali princìpi, non solo sono cogenti, ma sono princìpi di efficienza dell'economia pubblica e soprattutto princìpi fondamentali per riportare il nostro Paese a disporre di una pubblica amministrazione che sia motore e stimolo dello sviluppo economico e non soltanto un fattore di costi. Dicevamo che questa legge supera una giungla di disposizioni. Ricordo il testo unico degli impiegati del 1957, il n. 3, che aveva istituito il sistema delle carriere. nel 1980 fu approvata la legge n. 312, che istituiva i livelli retributivi ed i profili professionali. In seguito, abbiamo modificato il sistema di contrattazione collettiva con la legge n. 83 del 1993; siamo arrivati alla riforma ed alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e tuttavia la pubblica amministrazione continua ad essere ancora oggi considerata uno strumento di ritardo nell'erogazione dei servizi, ma soprattutto nell'espressione e nell'esercizio dell'attività autoritativa. Quindi, bene questa legge fa ad intervenire sull'attività provvedimentale, sull'esercizio e sul sul giudizio in merito alla responsabilità della pubblica amministrazione e dei pubblici dipendenti. L'introduzione, peraltro, della misura e dell'esercizio della *class action* costituisce uno strumento rafforzativo della tutela degli interessi legittimi dei cittadini e soprattutto fa sì che la posizione dei cittadini rispetto alla pubblica amministrazione sia totalmente diversa: infatti, tale tutela non costituisce più strumento derivato dell'attività provvedimentale, ma esercizio ed espressione di diritti fondamentali, di diritti civili. Dicevo, signor Ministro, che a questa riforma tuttavia manca un pezzo importante, che spero che prima della votazione di questo provvedimento si possa all'intervento su quel pezzo della pubblica amministrazione che costituisce l'unica funzione amministrativa costituzionalizzata esistente nel nostro Paese e cioè il complesso delle Forze di polizia e delle Forze armate. Lo voglio sottolineare qui, perché forse in quest'Aula mai era stato rilevato che l'unica funzione amministrativa costituzionalizzata è quella delle forze di polizia e delle Forze armate, citate nella prima parte della Costituzione negli articoli 13 e 17. Ebbene, questo importante plesso della pubblica amministrazione, che eroga servizi ed è in testa ai consensi dei cittadini italiani,

2004, la legge n. 350 del 2003, costituisca un ritardo che questa maggioranza, il PdL e l'attuale Governo debbano colmare. signor Ministro, in questo modo saremo in grado di applicare una riforma della pubblica amministrazione omogenea per settori, ma soprattutto per tipologia impiego e di funzioni. realtà, occorre dare ulteriore forza e corroborare tutte le iniziative legislative che hanno portato al decentramento amministrativo e, successivamente, agli interventi di attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso cui abbiamo modificato il sistema di ripartizione legislativo tra Stato e Regioni. Nell'applicare il federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, non possiamo lasciare indietro e da parte la riforma della pubblica amministrazione, che è strumento servente di tali leggi, ma soprattutto è strumento di efficienza della pubblica amministrazione attraverso la direttiva politica che parte dalle suddette leggi e che costituiscono il viatico fondamentale di riforme di cui l'Italia ha bisogno. Senza una pubblica amministrazione riformata, efficiente e produttiva non saremo in grado, pur nel contesto delle riforme che stiamo varando in Parlamento, di realizzare l'interesse pubblico diretto a dare maggiore soddisfazione ai bisogni pubblici e di ridurre contestualmente la spesa pubblica. Signor Ministro, onorevoli colleghi, signor Presidente,

dovremo vigilare attentamente sull'attuazione di questa riforma in sede di attuazione di decreti delegati. Quattro milioni e mezzo di dipendenti pubblici hanno infatti fiducia nell'attuazione di tale provvedimento e credo che dovremo dare un messaggio chiaro, che sarà quello di corroborare la produttività, l'efficienza alle dipendenze della pubblica amministrazione. Tuttavia, questo rapporto non potrà essere disgiunto, signor Ministro, da trattamenti retributivi più rispondenti alle prestazioni che saranno richieste ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il rapporto sinallagmatico tra le funzioni e le retribuzioni non può essere confinato nel ristretto ambito delle ristrettezze economiche pubbliche; il rapporto deve essere corretto e - lo ripeto - sinallagmatico, per far sì che le maggiori prestazioni richieste alle pubbliche amministrazioni siano poi effettivamente retribuite secondo canoni di ragionevolezza, di merito e di proporzionalità.

relatore*. Signor Presidente, devo ringraziare tutti gli onorevoli colleghi per la qualità dei loro interventi, i quali hanno confermato sino in fondo la straordinaria intensità per certi versi, persino la drammaticità dal punto di vista culturale della riforma che oggi il Senato si accinge a licenziare in materia di lavoro pubblico.

quasi di paura e di incertezza che in taluni interventi è stato colto, come se vi fosse una sorta di timore rispetto alla *mission* dell'innovazione. Ma credo che questo sia il tempo in cui debbano essere sottolineate le ragioni dell'unità, della convergenza e della confluenza, e non quelle della separazione. Pertanto, poiché sappiamo che riformismo è grande fatica, eluderò nella replica di sottolineare taluni tratti persino contradditori di alcune posizioni, soprattutto quando essi siano in qualche misura riferibili ad aree culturali che stanno manifestando renitenza al cambiamento, quel cambiamento che invece al Paese è è così necessario. la pubblica amministrazione si appresta ad avere squadernato di fronte a sé, da un lato uno scenario temporale lungo che non prevedrà la disponibilità se non di risorse significativamente inferiori per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, e dall'altro invece una domanda crescente, sempre più significativa e condensata di incremento della qualità, della tempestività e dell'efficacia nell'erogazione dei servizi ai cittadini clienti e utenti,

Se è così (ed è così), davvero viene in mente la frase di quel grande manager internazionale che, descrivendo la situazione del suo*business* - ma è anche quella della pubblica amministrazione - disse che bisognava cambiare il motore dell'aereo in volo,

noi quell'operazione, in sé audacissima e tecnicamente difficilissima, dobbiamo implementarla. È quello che questo disegno di legge fa: riscrive dalle fondamenta le regole di funzionamento della pubblica amministrazione. Quali sono i *driver* del cambiamento? Innanzitutto, si abbandona la tradizionale cultura del procedimento per passare alla cultura del provvedimento: ciò che misura infatti l'azione della pubblica amministrazione è la capacità dei suoi provvedimenti di intercettare la missione per la quale la struttura pubblica è stata istituita. Si trapassa da una pura cultura della neutralità della garanzia della guarentigia ad una cultura della capacità di incisione profonda della soddisfazione del bisogno pubblico per il quale la macchina è stata autorizzata ad esistere e a funzionare. È un cambiamento drammaticamente profondo, ma non potrebbe non avvenire, perché, mentre finché vige uno *status* *quo* tranquillo e persino pigro la cultura della garanzia ha una sua qualche ragione di esistenza e di buon funzionamento, in momenti di cambiamento così profondo, impegnativo ed essenziale per la possibilità stessa di sopravvivere della nostra Nazione, è evidente che bisogna avere la capacità di cambiare proprio l'atteggiamento antropologico con il quale la pubblica amministrazione funziona. Se questi dunque sono i tratti fondamentali del cambiamento, dobbiamo dire che vi è stata una grande capacità di coglierli fino in fondo in questo provvedimento che esce dalla confluenza di due proposte che hanno portato elementi di ricchezza al risultato finale.

sharing* e può essere erogata solo all'effettivo conseguimento dei risultati reali, misurati e certificati di miglioramento della produttività, della qualità e dell'efficienza della struttura affidata al dirigente. È una norma avanzatissima,

un possente *benchmark* di trasparenza e un vettore di modernizzazione anche per le aziende private. E quella paura paventata paventata da tante parti e da tanti segmenti dell'opposizione in ordine ad una sorta di rilegificazione non ha ragion d'essere, perché questo provvedimento - con una prospettiva culturale, federale e girondina - valorizza l'autonomia delle parti sociali e quella contrattuale, in cui la responsabilità delle parti sociali si materia, si invera e si realizza. Certo, lo fa con una dimensione dinamica - tipica dell'abbandono di un modello centralista ossessivamente burocratico, giustappunto giacobino - capace di modularsi in un'autentica, dispiegata prospettiva comunitaria. Una pubblica amministrazione comunitariamente attenta è la chiave di successo per questa stessa pubblica amministrazione.

*hindrance*, un elemento di affaticamento e appesantimento del nostro complessivo sistema competitivo, oggi si trasforma invece in uno strumento di accelerazione competitiva. Per la prima volta nella storia del Paese, con questo provvedimento la pubblica amministrazione è chiamata e vocata a diventare culturalmente titolare della *leadership* dell'innovazione. È una sfida alla quale, sono sicuro, nessun dipendente e nessun funzionario pubblico degni di questo nome avranno il coraggio di sottrarsi: torna tutta la nobiltà dell'espressione funzionario pubblico, in cui ciò che è pubblico - perché è comune, generale e collettivo - è più importante di ciò che invece ha soltanto

la pubblica amministrazione produce beni e servizi per 60 milioni di cittadini italiani: i salari dei 3,65 milioni di dipendenti pubblici ammontano a più di 190 miliardi di euro l'anno; della pubblica amministrazione, compresi quelli intermedi, è di quasi 300 miliardi di euro l'anno.

costi, ma non il giudizio della concorrenza. Quello che il professor Ichino chiamava *exit* e *voice*, cioè la possibilità di scegliere

Con questa riforma, non intendiamo privatizzare la produzione dei beni e dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, cosa difficile da fare, per la qualità dei beni in sé e che, nella storia anche recente, non sempre ha dato buoni risultati. Intendiamo semplicemente inserire elementi forti e fondanti di trasparenza, di giudizio, di valutazione e di soddisfazione dei clienti, nella produzione di tutti i beni e servizi pubblici. Trasparenza (*exit*) vale a dire avere la possibilità di spostarsi da una produzione all'altra di questi beni e servizi pubblici

chiara e forte, con le relative conseguenze, la propria voce (soddisfazione dei clienti, *in primis*). Non li chiamo più utenti, li chiamo clienti: i 60 milioni di cittadini italiani sono dei clienti, non sono degli utenti. Il disegno, onorevoli colleghi, è semplice. Non aggiungo molto altro. L'Italia, il Paese è maturo per questa riforma. Lo chiede la gente, lo chiede l'Unione europea, lo chiede il nostro tasso di crescita che è strutturalmente basso nei confronti dell'Unione europea, al di là delle crisi, proprio perché la competizione, dopo la moneta unica, si fa sull'efficienza del sistema e il sistema, in gran parte, è dato dalla nostra pubblica amministrazione: una pubblica amministrazione inefficiente

di chi ha più bisogno, è l'Italia dei più deboli a chiedere una pubblica amministrazione efficiente, una pubblica amministrazione di qualità, una pubblica amministrazione gentile consapevole di essere una risorsa fondamentale per il Paese, quando è efficiente; ma una palla al piede quando è inefficiente, opaca, insensibile ai bisogni della gente. Questa è una riforma per lo sviluppo del nostro Paese, per avere più efficienza, più giustizia, più equità. Per questo, colleghi, ho voluto fin dall'inizio dell'*iter* di questo provvedimento ascoltare con

parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.323, 5.301, 3.324, 7.305 e 7.304. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.305 e parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

semplice. Questo emendamento si propone di scongiurare il rischio che compaia nel testo il principio di regionalizzazione del concorso pubblico. Non siamo d'accordo con l'idea che in Lombardia ci debbano essere solo professori lombardi e in Calabria solo professori calabresi. Preferiamo la mescolanza dei generi e delle culture.

Sono tutti emendamenti che trattano la questione della regionalizzazione dei concorsi, tema che è diventato particolarmente di attualità anche in relazione al dibattito sulla scuola. Anzitutto ci sono problemi di costituzionalità a questo proposito, ma non è questo che mi interessa sottolineare nel motivare

lo spirito che muoverebbe questo

Il problema è che in tutti i concorsi pubblici ci si presenta da tutt'Italia, vincono i concorsi magari persone che provengono da altre Regioni; vivere a Milano, appena hanno la minima possibilità legislativa, chiedono il trasferimento per tornare nella

perché i nostri giovani non partecipano ai concorsi. Forse con l'aria che tira probabilmente cambierà anche questo, non partecipano ai concorsi per gli stipendi da fame della pubblica amministrazione. Mi spiace aver sentito il Ministro ricordare soltanto il costo globale della pubblica amministrazione e non anche gli stipendi medi dei suoi dipendenti. Allora, se vogliamo

ai nostri ragazzi anche culturalmente, bisogna sapere che si deve agire sugli incentivi economici perché altrimenti i giovani milanesi o lombardi neolaureati non andranno a

1.18 e 1.305

abbia espresso un parere contrario. Ciò mi sembra irrituale e, vorrei dire senza offesa, vergognoso. Mi rendo conto che non tutti hanno interesse ad ascoltare;

corposa del 30 per cento delle spese, a volte inutili, al servizio di elefantiaci uffici che servono soltanto per dare ulteriori prebende e non a migliorare il rapporto tra il cittadino

sensibile. Mi appello al Governo e al relatore perché prima di passare al voto vi sia un ripensamento forte e non indifferente,

circostanza che questo è già stato fatto per gli uffici di diretta collaborazione con i regolamenti *ex* comma 404 e seguenti della legge finanziaria del 2007 per la Presidenza del Consiglio dei ministri è avvenuto all'inizio della legislatura in corso. Mi rendo conto che si è sempre popolari quando si fa un discorso di ridimensionamento delle spese perché ci sono uffici elefantiaci,

in corso. So che il ragionamento del senatore Cintola è sicuramente molto più popolare del mio, ma personalmente mi attengo anche alle regole di una pubblica amministrazione che non deve avere troppo ma non deve avere neanche troppo poco.

perché se in un momento di crisi così grave siamo tutti costretti a fare i conti con la riduzione della spesa pubblica, non capisco perché tagliamo in settori vitali e non possiamo ulteriormente ridimensionare - naturalmente non con populismo, ma con accortezza ed intelligenza - anche le strutture di diretta collaborazione. Poiché nell'emendamento c'è un preciso riferimento alla misura del 10

agli atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti in questo periodo appare fuori questione. L'emendamento 2.304

propone di sostituire le parole «per la fissazione di vincoli alla» con le parole «di regolazione della», perché si vuole prevedere che vengano individuati semplicemente i criteri di regolazione della contrattazione collettiva, e non invece i criteri di fissazione di vincoli alla stessa. È un tema che ho trattato esplicitamente nel mio intervento in discussione generale, nel provvedimento in esame, si cercava di trasferire competenze dalla contrattazione alla legislazione, individuando nella legislazione i criteri per fissare i vincoli alla contrattazione medesima. L'emendamento è volto ad affermare il principio per cui i decreti delegati, nell'individuazione dei criteri di regolazione della contrattazione collettiva integrativa, al fine di rispettare i vincoli di bilancio, debbano assicurare, allo stesso tempo, adeguate garanzie e tutele nei confronti del lavoratore, nelle ipotesi di assenza per causa di malattia o di infortunio contratto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

lettera *e)*, cioè la disposizione secondo cui si prevede che vengano individuati, non semplicemente i criteri di regolazione,

L'emendamento 2.305 riguarda l'argomento trattato all'inizio del mio intervento in Aula, a proposito della commistione poco convincente tra spirito del settore privato e spirito del settore pubblico. Si cerca di evitare che il riordino delle procedure di contrattazione collettiva avvenga secondo metodi cosiddetti prevalenti all'interno del settore privato.

dire, su una logica di tipo sintattico: non si capisce come si possa esercitare un controllo su un periodo di tempo successivo allo svolgimento dell'incarico di componenti delle organizzazioni sindacali.

diverso rispetto a quello del disegno di legge a proposito del rapporto fra settore privato e settore pubblico. la pubblica amministrazione abbia e/o debba avere valori di riferimento diversi rispetto a quelli di un investitore privato: si suppone che quest'ultimo sia interessato, prima ancora che al bene comune, all'efficacia dei propri affari, mentre al settore pubblico il cittadino deve chiedere servizi

Commissione ha chiarito in maniera più precisa del testo originale la questione relativa alle materie del contratto e della legge, però, anche sentendo il senatore Castro,

affermazioni condivisibili sulla separazione tra legge e contratto, sarei per togliere ogni dubbio. Sarebbe anche un segno

specificità pubbliche che in terreno contrattuale, proprio dopo la privatizzazione del rapporto del lavoro, in realtà non ci devono essere. Per evitare cose di questo genere chiedo al Ministro

dichiarazione di voto. applicare nel settore dell'impiego pubblico una norma generale di diritto comune che si applica ai contratti di diritto privato. Sopprimerla va in senso contrario alla logica generale dell'ordinamento.

con l'emendamento 2.303 vorremmo fissare vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio. Signora Signora Presidente, onorevoli colleghi e signor Ministro, ho sentito parlare in quest'Aula da valenti colleghi della *class action* nella pubblica amministrazione; peccato che quella *class action*, che doveva entrare in vigore il 1° luglio per tutelare i consumatori ed il mercato, sia stata rinviata alle calende greche; non solo, essa è stata svuotata di qualsiasi contenuto. Abbiamo i risparmiatori truffati della Parmalat, della Cirio e dei *bond* argentini che aspettano ancora giustizia

abbiamo la maggioranza di questo Governo che parla di *class action* nella pubblica amministrazione non rendendosi conto del danno che arreca al mercato, perché scrive i suoi rinvii sotto diretta dettatura delle banche e della Confindustria. Per

il nostro Gruppo voterà contro questo emendamento, perché pensiamo che l'unificazione pubblico-privato sia stato un elemento di chiarezza, importante per i lavoratori e di trasparenza per i cittadini, quindi non capiamo questo riproporre delle specificità.

Sappiamo che già dal decreto legislativo n. 29 del 1993 in poi questo è stato un elemento molto forte di innovazione del settore privato. Tante cose non sono andate bene, su di esse riflettiamo, ma sicuramente tornare indietro in questa direzione non ci convince, pertanto voteremo negativamente.

Sono episodi veramente deleteri. Mi auguro che ciò non si ripeta, ma posso solo ricordare ai senatori che il voto è un diritto fondamentale e importante nell'esercizio del proprio mandato e sarebbe bene usarlo correttamente.

dei rapporti tra le fonti, cioè tra la contrattazione e la legge. Abbiamo cambiato un'impostazione viziata della proposta originale del Governo: non si riforma la pubblica amministrazione con botte di leggi, o peggio di leggine, ma valorizzando la contrattazione collettiva. Questo è un punto fondamentale. Abbiamo migliorato e introdotto princìpi virtuosi su quattro punti fondamentali che vorrei ricordare: il chiarimento del ruolo importante della contrattazione e quindi della responsabilità sociale per migliorare il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; la semplificazione del procedimento amministrativo che è decisivo per ottenere i risultati ed è un punto stranamente dimenticato dal Governo;

la valorizzazione dei rapporti con le autonomie anche nell'attuazione della delega, che è sempre un procedimento complicato. Abbiamo infatti coinvolto la Conferenza unificata perché sia garantita l'attuazione precisa

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 847, impegna il Governo a porre in essere misure di ridimensionamento e razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti negli uffici di diretta collaborazione, provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture

secondo le procedure ordinarie e tenderà a realizzare una riduzione della spesa per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni.

finale, perché anche qui il lavoro che abbiamo fatto ha reso chiaro il principio della convergenza tra sistema pubblico e gestione privata dei rapporti di lavoro.

Colleghi senatori, per favore, un attimo di calma: stiamo procedendo bene, però abbassate la voce. di un combinato disposto volto a favorire l'individuazione e la rimozione, da parte degli organi di valutazione indipendente, delle situazioni di grave sofferenza sul piano dell'efficienza e della produttività delle amministrazioni.

nel provvedimento a danno delle società concessionarie quotate o in cui un soggetto pubblico detiene quote minoritarie, così come per le società prevalentemente partecipate non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Aggiungere la *class action* delle pubbliche amministrazioni comporterebbe, a mio parere, un aggravio dei costi di gestione, l'incremento dei rischi connessi e criticità legate all'incertezza del quadro di riferimento, nonché un difficile coordinamento delle relative discipline (privatistica e pubblicistica) che avranno procedure distinte. Occorre, in primo luogo, sottolineare che le società quotate e quelle da esse direttamente partecipate operano in conformità con le regole di mercato che impongono loro di creare valore

diversi operatori alla ricerca della massima efficienza e qualità del servizio prestato a beneficio degli utenti finali. Per tali caratteristiche e per il fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, le società quotate, anche nelle ipotesi in cui siano concessionari di servizi pubblici, non possono essere equiparate alla pubblica amministrazione. Ugualmente, tale equiparazione non ha ragion d'essere nei confronti di quelle società in cui un soggetto pubblico detenga una partecipazione inferiore alla metà del capitale sociale. Queste ultime, pur essendo concessionarie di servizi pubblici, operano come società private e come tali - come già ricordato - sono già assoggettate alla disciplina della *class action* privatistica, di cui al codice di consumo. Tale interpretazione risulta coerente, tra l'altro, con la recente revisione della disciplina per la responsabilità per danno erariale che ha circoscritto l'ambito di intervento della Corte dei conti e la conseguente configurazione di ipotesi di danno erariale in capo agli amministratori delle pubbliche amministrazioni e delle società in cui lo Stato detenga più del 50 per cento del capitale sociale. Indiscutibilmente anche le società prevalentemente partecipate non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione operano in conformità delle regole di mercato e come tali sono già assoggettate alla disciplina della *class action* privatistica, di cui al codice di consumo. Tali società, infatti, conseguono, tra l'altro, ricavi da mercato e il *management* è dotato di ampia autonomia alla stregua del *management* di un'azienda di tipo *market*, con conseguente esposizione alle In conclusione, la scelta di equiparare alla pubblica amministrazione i concessionari di pubblici servizi, indistintamente dalla reale partecipazione azionaria dello Stato, dalla loro quotazione in Borsa ovvero dal non far parte delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, rischia di determinare ambiguità e confusione nell'ambito di applicazione e nel concreto esercizio dello strumento della *class action* da parte degli utenti finali. Per tale motivo è necessario operare una netta distinzione, in termini di ambito applicativo, tra le due fattispecie di azione collettiva, escludendo dall'ambito di applicazione del provvedimento in discussione le società quotate in Borsa, le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale, ovvero le società prevalentemente partecipate non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione operano

perché, oltre ad appartenere alla nostra cultura di riforma della pubblica amministrazione, è anche presente in molte buone prassi di alcune nostre amministrazioni

istituire un'agenzia di valutazione, però ci rende perplessi la stima della spesa di questo nuovo organismo, il cui costo ammonta a 4 milioni di euro per il 2009 e a 8 milioni di euro per il 2010.

a prevedere che i componenti del nuovo organismo non siano superiori a cinque, ma soprattutto che prestino la loro collaborazione a titolo gratuito, e ancora che siano scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, perché rivestono incarichi elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o perché intrattengono rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con tali organizzazioni. Detto in maniera più esplicita, si ritiene che, nella costruzione di questa agenzia di valutazione, si debba sorvegliare nel modo più rigoroso per evitare la costituzione di conflitti di interesse.

lo dovessero ritenere il relatore e il Ministro, eventualmente di trasformare questo emendamento in un ordine giorno per suggerire suggerire di comunicare in tempo utile ed opportuno gli obiettivi da raggiungere in modo da velocizzare l'azione dei dirigenti e quindi renderla più efficace ed efficiente rispetto all'obiettivo che la stessa amministrazione si dà.

nei tempi e nei modi per evitare sovrapposizioni inutili. Ovviamente, l'azione collettiva risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, soprattutto quando riguarda le carte dei servizi,

Il contenuto delle due disposizioni è sostanzialmente lo stesso.

3.323 e 3.325, in quanto sopprimono la copertura finanziaria dell'organismo di valutazione; 3.324, perché modifica quella copertura finanziaria,

Il parere contrario è stato espresso sul presupposto che si tratti di una mera ripetizione del principio di trasparenza che noi abbiamo effettivamente enunciato. Faccio presente, però, che

dei dati sui quali gli organi di valutazione svolgeranno la loro attività di misurazione, valutazione ed elaborazione degli indici di andamento gestionale. L'emendamento 3.326 mira ad ampliare

si estende il principio di trasparenza a tutti i dati relativi al funzionamento dell'amministrazione pubblica, salvo ovviamente quelli qualificati come riservati. Non esiste alcun principio che possa giustificare l'occultamento di qualcosa che accade nel settore pubblico, salvo si tratti di evento riservato, qualificato come tale. come tale. Se vogliamo allinearci con il meglio delle esperienze nordeuropee, dobbiamo compiere questo piccolo passo in più, quello che ci separa

Signora Presidente, ho ascoltato attentamente le ulteriori spiegazioni fornite dal senatore Ichino. Poiché la trasparenza rappresenta uno degli elementi che hanno caratterizzato

su punti di merito non necessariamente sempre lo stesso schema di maggioranza e opposizione, altrimenti la nostra funzione sarebbe completamente alterata.

La norma che introducete, infatti, relativa alle modalità di valutazione dei sistemi dell'amministrazione, che è quella del *benchmarking*, cioè delle valutazioni territoriali,

attraverso il confronto dei risultati e dei livelli di efficienza raggiunti (e quindi arrivando a far costruire dalle amministrazioni medesime gli standard qualitativi per il confronto stesso) i modi per rendere la valutazione non burocratica e punitiva, ma efficiente, premiale e quindi capace di innescare meccanismi virtuosi.

che invece noi abbiamo proposto e sulla quale ci siamo molto battuti, che attiene all'Agenzia per la valutazione, agli standard previsti dall'Agenzia e quindi al sistema di terzietà e di qualità che noi vogliamo introdurre nella pubblica amministrazione rispetto al tema della valutazione. Si sa infatti che molto spesso gli schemi della valutazione sono saltati perché troppo poco qualificati o troppo dipendenti dalla politica. Invece, l'elemento della terzietà, della competenza e della qualificazione è quello che assicura davvero un processo trasparente di valutazione e di competenze.

«indipendenza e autonomia» può apparire una endiadi, ma l'indipendenza è la caratteristica che abbiamo voluto imprimere all'intero sistema di valutazione con una disposizione riguardante l'Agenzia centrale, che prevede la nomina del vertice dell'Agenzia con il consenso di due terzi del Parlamento. Tale consenso mira proprio a sottolineare l'indipendenza dell'Agenzia centrale dal potere politico e la stessa indipendenza deve realizzarsi ai livelli inferiori rispetto ai livelli inferiori del potere politico. Voi potreste dire che la parola «autonomia» già comprende questo concetto, ma a me sembra che rafforzarlo vada nella stessa direzione dell'intero disegno di legge.

E non abbiamo nemmeno compreso, a dire il vero, a meno che il relatore non ce lo spieghi (per cui possiamo anche rivedere la nostra opinione), il motivo del parere contrario, richiamandosi questo, se non abbiamo capito male, al coordinamento di alcuni testi relativi alle azioni collettive, che peraltro hanno fatto parte di una serie di nostre proposte. Vorremmo pertanto capire nel merito, se fosse possibile, la motivazione

dalla senatrice Incostante,

e naturalmente siamo molto soddisfatti che lo stesso verrà accolto. Mi sembra che l'aver introdotto la trasparenza come uno dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni sia un grande passo avanti di cultura politica, giuridica e speriamo anche di concreta vita delle nostre pubbliche amministrazioni. Naturalmente, le norme sono importanti e noi ci siamo battuti per questo, ma siamo convinti che se non si innescherà un'azione, vera e di lungo corso, di reingegnerizzazione dei processi e di premialità nella riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche questi sforzi notevoli che avremo compiuto non potranno arrivare a risultati significativi. Quindi, come vedete, continuiamo ad essere molto impegnati su questo tema ed a sfidare il Governo

Presidente, vorremmo sottolineare il valore, che non è enfatico qualificare come storico, di questa norma che stiamo per approvare, perché non soltanto con essa ci allineiamo con i due ordinamenti più civili e avanzati d'Europa sul terreno della trasparenza totale delle amministrazioni pubbliche, ma combiniamo il principio di trasparenza con il principio di valutazione, in un rapporto di sostegno reciproco. La valutazione acquisterà

di svolgere la valutazione sulla base degli stessi dati e di confrontare la valutazione espressa dagli osservatori qualificati, ricercatori universitari, associazioni di utenti, stampa specializzata, con quella del

i più avanzati ed efficienti su questo terreno. E non è tutto: la trasparenza della valutazione e il coordinamento che l'agenzia centrale imporrà al fine di rendere confrontabili gli indici di andamento gestionale di tutte le tutte le amministrazioni fra loro omologhe consentirà ai cittadini di vedere inserite in una graduatoria di efficienza e produttività tutte le amministrazioni e tutti i servizi. Finalmente potremo sapere se l'ospedale della nostra Provincia o del nostro quartiere rende servizi simili, migliori o peggiori rispetto a tutti gli altri ospedali; potremo valutare comparativamente l'efficienza delle nostre polizie locali, delle nostre scuole, dei nostri servizi di formazione professionale e così via. via. Ciò consentirà, finalmente, anche di imporre alla dirigenza pubblica obiettivi precisi, misurabili e quindi cogenti ai quali agganciare non soltanto il premio per il risultato

Con compiacimento mi sento di dire che nel settore dell'università il principio della trasparenza è già stato introdotto concretamente nel nostro sistema giuridico.

di un sistema premiale che è quello che poi qualifica nei migliori sistemi privati l'efficacia della valutazione e del funzionamento delle risorse umane. stabiliti con precisione, dunque non genericamente, gli obiettivi di valorizzazione del merito, vale a dire quante risorse devono essere dedicate, il fatto che ciò significhi più selettività anche nelle carriere,

efficacia ed efficienza. Quindi, non vorrei dilungarmi, ma sottolineo che anche per noi questo è un risultato positivo e di miglioramento di una norma che era nata un po' storta, ma che alla fine è

l'atto di indirizzo che il ministro Sacconi ha inviato alle strutture sanitarie di tutte le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, Trento e Bolzano, che sta producendo una dolorosa sospensione di una scelta fatta dal tutore della famiglia Englaro e sancita da una sentenza della Cassazione e da un parere della Corte costituzionale.

«Stato vegetativo e stato di minima coscienza» del novembre 2008 che parla di stati vegetativi non permanenti, ma persistenti, definiti «potenzialmente reversibili»

e, personalmente, lo considero un modo surrettizio di riproporre un conflitto di attribuzione con la Cassazione già respinto dalla Corte costituzionale. È un atto tra il pilatesco e l'azzeccagarbugli per non affrontare un problema che va affrontato in questa sede, non dal Governo, ma dal libero gioco di maggioranze e minoranze, entrambe libere seconda coscienza.

che la crisi mondiale fondata sulle piramidi finanziarie che sta devastando l'economia, falcidiando posti di lavoro, bruciando i risparmi di milioni di famiglie, meriti attenzione. Mi riferisco, per esempio, al

che riguarda le famiglie, il risparmio e le imprese (soprattutto quelle piccole e medie) che,

nuova finestra") tecnicamente inutile perché, se fossimo in diritto amministrativo, diremmo che è cessata la materia del contendere, che era stata presentata un mese e mezzo fa, sugli orari ferroviari per i pendolari. L'orario è entrato in vigore domenica il Governo non ha ancora risposto: le ferrovie non l'hanno quindi cambiato e i pendolari stanno pagando il prezzo di quest'assurda modalità che il Governo ha di gestire il rapporto con i propri cittadini governati. di fronte ad un'assoluta volontà di non rispondere alle interrogazioni del Parlamento, o i parlamentari dovranno compiere le classiche azioni per le quali finiscono sulle pagine dei giornali, in modo tale da attirare l'attenzione, oppure penso sia inutile stare in questo Parlamento, perché tanto il Governo non risponde alle prerogative dei parlamentari. Mi appello alla sua capacità di intervenire presso il Consiglio di Presidenza perché il pregio di questo Senato sia rispettato. Comincio a dubitare che anche il Consiglio di Presidenza sia in grado di ottenere dal Governo una risposta, visto che mi risulta - e non ho motivo di pensare il contrario - che più e più volte sia stato sollecitato l'Esecutivo, nel nome dei Ministri competenti (e cioè quello dell'economia e quello dei trasporti), a rispondere in questa sede, ma ciò non è avvenuto. Ne dobbiamo prendere atto? No, mi rifiuto di farlo: e allora, ogni volta prenderò la parola per protestare formalmente perché il Governo non risponde a queste interrogazioni. E siccome qualche collega gode di questo tipo di atteggiamento, segnalo che i primi a rimetterci sono proprio i loro elettori. Non è un problema di bandiera, ma di rispetto delle prerogative del Parlamento e, prima di tutto, di quelle dei cittadini. Senatore Lusi, le do la stessa risposta che ho già avuto l'onore di darle tempo fa, e cioè che questa Presidenza ha più volte sollecitato il Governo,

dando il via ad un'iniziativa molto ragionevole e sensata, riconoscendo che l'accanimento terapeutico è una cosa, l'alimentazione e l'idratazione un'altra. Si tratta di due cose distinte e molto diverse

al di là dell'evocazione natalizia del collega Leoni, c'è un profilo molto più forte che emerge dal provvedimento di cui discutiamo.

si dice come il diritto alla nutrizione e all'idratazione abbia un profilo di tutela e di garanzia irrinunciabile. Certo, mi rendo conto dei richiami che sono stati fatti al drammatico caso di Eluana Englaro, ma proprio da quando abbiamo cominciato in Cassazione e poi in Parlamento - a discutere del caso di Eluana Englaro nel mondo dei disabili si è diffusa un'ansia, un'angoscia, quantomeno una preoccupazione che richiedeva, dal mio punto di vista, giusta e doverosa presa di posizione da parte del Ministro. Non dimentichiamo che fra le ragioni per le quali il Ministero della sanità, che era stato abrogato in una consultazione referendaria, è stato risuscitato vi è questo profilo

Presidente, ha ragione. Non avevo alcuna intenzione di intervenire. Mi sono trattenuto per puro caso in Aula e sono stato costretto a sentire delle cose inverosimili di fronte alle quali devo esprimere una mia opinione. Trovo assolutamente pazzesca la presa di posizione del ministro Sacconi: è un tentativo surrettizio di replicare un contrasto che è già stato risolto.

con meno di dieci righe di motivazione, perché non ne meritava di più, e la questione è stata chiusa. La Corte costituzionale ha dato ragione alla Corte di cassazione, che a sua volta aveva dato ragione al tribunale. La storia di questa povera persona non trova una fine e adesso dobbiamo assistere a questa retorica questa retorica insopportabile per cui un Ministro adotta un provvedimento amministrativo contro le decisioni della giustizia per costruire, per l'ennesima volta, una falsa e orribile polemica per cui il centrodestra sta dalla parte della vita e il centrosinistra dalla parte della morte. Sono allibito, costernato e avvilito Senatore Gramazio,

le varie parti politiche - ad una sorta di campionato di serie B, in cui sostanzialmente affrontiamo le tematiche, che molto spesso dovrebbero essere prerogativa del Parlamento, in una sorta di girone di ritorno. Allora, torno ad insistere

La collega Silvana Amati ha presentato un disegno di legge in merito, che hanno firmato colleghi di destra e di sinistra; lo stesso Ministro degli affari esteri, come commissario europeo, ha proclamato una giornata contro la tratta l'anno scorso. Non ho motivo di ritenere che ci sia qualcuno contrario; c'è un ritardo della politica ad affrontare questo problema mentre continuiamo a parlare di sicurezza

in questo Paese, possa portare avanti il proprio lavoro in tempi certi, ma allo stesso tempo che alcuni argomenti possano diventare come iniziativa parlamentare un momento di confronto, non solo tra i soliti dieci.

un dibattito più ampio, anche perché ricordo che, con il voto contrario della delegazione radicale, a fine luglio è stato adottato un ordine del giorno in cui si includeva includeva all'interno dei nostri lavori il dibattito relativamente al testamento biologico. Ebbene ad oggi tutto ciò non è arrivato. Mancano sì e no tre o quattro giorni di lavoro, nella migliore o nella peggiore delle ipotesi (a seconda dei gusti) e quindi non credo che arriveremo a dibattere di tutto questo. Il senatore Gramazio ha avuto l'ardire di affermare che i giudici ancora una volta si sono infilati nella dinamica che dovrebbe regolamentare la vita e la morte. però i giudici non lo possono fare, non si riesce a capire il motivo per cui un esponente del Governo lo possa fare. Se si parla di diritto, sicuramente non si deve parlare di dovere; altrimenti trascorreremo le feste natalizie con una serie di trattamenti sanitari obbligatori che rovineranno - quelli sì - le feste di molti italiani! [MARINO

Credo sia abbastanza sorprendente che ci si preoccupi di una convenzione del 13 dicembre 2006 quando non si è ancora depositato lo strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, che richiede semplicemente - lei, signora Presidente, lo sa molto meglio di me - che qualcuno del Governo si rechi nelle sedi appropriate e depositi fisicamente la ratifica della Convenzione.